Signor Presidente, onorevoli colleghi, sento il dovere di prendere la parola a titolo personale. Voltaire diceva: «Ama la verità e perdona l'errore». E proprio l'accostamento di verità ed errore è la metafora di un percorso che mi ha visto protagonista negli ultimi tre anni. anni. Esattamente tre anni fa si diffondeva, infatti, la notizia di un'indagine della procura di Roma su presunte truffe all'INPS nella quale sarei stato coinvolto. Ovviamente il processo mediatico pronunciava la sua sentenza ben prima di qualsiasi dibattimento o raccolta di prove. Malgrado l'amarezza di un tale scenario e la conseguente sovraesposizione mediatica, ho deciso di amare la verità attendendo fiducioso l'esito delle indagini, mettendomi sempre e comunque a disposizione degli inquirenti, certo della totale estraneità dai fatti contestati. In questa stessa Aula, a poche ore dalla diffusione delle prime notizie, ho voluto metterci la faccia, dichiarando apertamente di rinunciare a ogni forma di immunità parlamentare, mettendomi a disposizione, senza filtri istituzionali, consegnando la mia dignità nelle mani della magistratura. In tre anni ha preso forma un percorso di verità che si è concluso con l'archiviazione disposta dal GIP il 7 giugno scorso, senza quindi che sia mai iniziato un processo; un'archiviazione che ha concluso un carosello di notizie infondate, di speculazioni giornalistiche e politiche che hanno superato il seppur legittimo diritto di cronaca. Ho voluto condividere con voi la risoluzione di questa vicenda, non per mero compiacimento o per semplice completezza di informazione, ma innanzi tutto per il rispetto che porto a quest'Assemblea e per fare della mia esperienza, che accomuna molti di noi, una testimonianza che sia monito ed esempio al tempo stesso; un monito verso chi ha l'ingenuità di credere che la verità sia quella urlata dai titoli di giornali; un esempio per chi crede che la verità, amata e ricercata, prima o poi arriva, malgrado il percorso incerto e complesso. Non voglio additare - prestando il fianco al facile populismo - le evidenti falle di un sistema in cui alla ricerca della verità talvolta si predilige dare priorità al clamore mediatico; sarebbe troppo semplice farlo in questo momento. Il mio è un invito alla riflessione e alla razionalità. Le gogne fanno male alla politica e all'Italia. Le dita puntate e le accuse urlate affossano il Paese, e in questo particolare momento storico nulla appare più evidente di ciò, oggi più che mai. Grazie ancora a chi mi è stato vicino e non ha mai dubitato di me.

luce delle diverse sentenze di primo grado dei tribunali dei minorenni, venisse risolta dalle sezioni unite della Cassazione affinché decidessero in maniera univoca quale interpretazione dare alla normativa vigente. Il procuratore della Repubblica, l'8 aprile, ci ha risposto con una cortese lettera, ci ha risposto con una cortese lettera, in cui si faceva carico delle nostre preoccupazioni, e ci assicurava che il 26 maggio, arrivando in Cassazione un ricorso su uno di questi casi, la procura si sarebbe costituita per fare chiarezza. la procura si è costituita, Presidente, e ha scritto testualmente che la procura generale chiede di rimettere alle sezioni unite la decisione in quanto si tratta di una questione della massima importanza su cui tutta l'Italia si interroga e su cui stanno indagando filosofi e psicologi, su cui il Parlamento sta riflettendo, avendo stralciato la *stepchild adoption* dalla legge Cirinnà. In questi casi scrive la procura generale della Repubblica - l'ordinamento affida la decisione alle sezioni unite, vertice deputato a porre le colonne fondamentali della giurisprudenza. Aggiunge, poi, la procura che solo le sezioni unite possono evitare che in Italia si determini una situazione "a macchia di leopardo" con decisioni diverse da Venezia a Messina; diversamente ogni giudice di merito darebbe la sua interpretazione. Questo ha scritto la procura generale. Ebbene, la prima sezione della Cassazione il 26 maggio ha già deliberato, ignorando totalmente l'appello della procura generale. Ha deliberato nel merito - vedremo come - e ieri ha deliberato di nuovo. Ricordo, Presidente, che la prima sezione avrebbe dovuto essere presieduta dal dottor Fabrizio Forte, che aveva i meriti di anzianità,

Abbiamo avuto dunque queste dimissioni clamorose. Non ci sono precedenti di chi, per anzianità e titoli, viene pretermesso. Il problema che pongo e che abbiamo di nuovo proposto al primo presidente della Corte di cassazione è questo ordinamento, anche ai massimi livelli, rispetta le regole? E le regole non sono quelle delle sezioni unite? E perché un problema così importante non va alle sezioni unite, visto che il Parlamento in qualche modo ha chiesto alla magistratura di fare chiarezza? Non vorrei che fossimo di fronte - lo dico al Presidente - all'ennesimo scardinamento, all'ennesimo esempio di ciò che Pannella chiamava "furto di legalità". È giusto stare alle regole. Noi accetteremo quello che le sezioni unite della Cassazione diranno, ma non accetteremo scorciatoie che umiliano il Parlamento e la volontà popolare.

Mi sembra che ci troviamo di fronte a una situazione che dovrebbe interessare l'intero Parlamento. Noi solleviamo il problema al Senato, e io sono uno dei firmatari delle richieste che il senatore Giovanardi ha brevemente illustrato. Il nostro è un intervento a difesa della legge, Presidente, per evitare che un provvedimento così controverso e discusso, ma alla fine approvato dal Parlamento, in una formulazione che il Parlamento ha ritenuto conforme alla propria volontà, possa trovare applicazioni diverse o addirittura opposte

il provvedimento è diventato legge dello Stato, credo sia interesse di tutti, delle istituzioni innanzitutto e del Parlamento della Repubblica *in primis*, fare in modo che essa sia rispettata nella sua integralità e non ci possano essere sentenze fantasiose o addirittura opposte. Pertanto, signor Presidente, le saremmo veramente molto grati se la Presidenza del Senato si interessasse di questo caso e ne informasse l'Assemblea.

Signor Presidente, ho preso atto delle proposte che ieri ha avanzato il vice ministro Zanetti. Per quanto riguarda la riformulazione che egli ci ha proposto, ritengo che in quei termini essa non sia accettabile, perché il tema di fondo è la durata di un'eventuale proroga delle concessioni in un Paese che ha concesso alle autostrade - lo dico per coloro che si scandalizzano

al vice ministro Zanetti se volesse valutare una riformulazione della riformulazione, nei termini seguenti: «a prevedere, tenuto conto degli investimenti immobiliari e infrastrutturali già effettuati, dei beni aziendali e delle professionalità acquisite in tutti questi anni, in relazione alle suddette novazioni, una proroga di trent'anni

senatore Gasparri per la sua controproposta, ma il Governo non è intenzionato a vincolarsi in questa sede a una specifica di un periodo transitorio, che è fermamente determinato a introdurre e altrettanto fermamente determinato a fare in modo che sia rispetto non certo solo a logiche di sistema, di normativa, di quadratura nazionale e comunitaria, ma ovviamente anche alle esigenze operative di chi lavora nel settore e di chi ha fatto investimenti. termine "adeguato" c'è tutta l'attenzione del Governo su questi temi e tutta la disponibilità a confrontarsi poi con il Parlamento nella costruzione della futura normativa. Riteniamo che in detta sede sia questo il modo giusto di affrontare la questione e, quindi, riconfermo la disponibilità alle riformulazioni proposte ieri. In alternativa il parere del Governo è contrario.

potrebbe essere riassumibile nello stato del procedimento ancora pendente davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, vale a dire tutto ciò che viene dopo la direttiva 2006/123/CE

ostare a una normativa nazionale di proroga. Pur tuttavia, il legislatore e il Governo italiani hanno fatto ben poco, subendo tutto tutto ciò che è conseguito alla comunicazione di infrazione e assumendo un atteggiamento di particolare inerzia, rotto solo da quelle proroghe - di cui si è parlato nei vari interventi - che hanno rappresentato ben poco per imprese che, comunque, devono fare i conti con una prospettiva temporale e di progetto economico della loro sostenibilità che non può essere

che avrebbero dato un assetto un po' più organico a tutta la questione dal punto di vista non solo del demanio, ma anche urbanistico e di uso del territorio *tout court*. Ebbene, nonostante questo e al di là degli errori, dei torti e delle ragioni,

applicare da subito la cosiddetta "direttiva Bolkestein" per le nuove concessioni), consenta di pensare a un regime di proroga che tenga conto non solo degli investimenti svolti, ma soprattutto

di un termine di una particolare prudenza, che serve semplicemente a portare a conclusione il percorso di un'impresa di tipo familiare,

Prendo atto che il Governo ha in parte dato la garanzia di portare a soluzione la questione. Forse avrebbe dovuto far molto di più per quanto riguarda il

Signor Presidente, dirò poche parole perché ieri, nel dibattito per la presentazione delle mozioni, abbiamo espresso chiaramente le nostre

che, insieme con le forze sindacali e sociali, lanciarono l'allarme sulla pericolosità dell'approvazione di quella direttiva europea, furono tacciati, ancora una volta, di essere ideologici

Ma anche quella fu una occasione per tacciare alcuni di noi come i soliti di sinistra che volevano radicalizzare e che si preoccupavano di chiudere il mercato. In realtà, quella direttiva, che si presentava come un'occasione per diminuire la burocrazia e i vincoli alla competitività nei servizi per il mercato interno,

quella famosa direttiva, da tanti osannata, avrebbe avuto impatti anche in importanti settori della nostra economia. Per questo oggi ci ritroviamo con una realtà

Noi pensiamo che la revisione di tutto questo possa essere anche l'occasione per rivedere la normativa, ad esempio, per garantire ai cittadini il libero accesso alle spiagge e la fruizione delle stesse. Ieri veniva ricordato nel dibattito che le spiagge libere di fatto non esistono più, e di questo gli enti locali dovrebbero farsi carico.

sia stato quanto meno singolare avere iniziato a parlare di concessioni demaniali a partire dalla mozione che ha presentato il senatore Gasparri giusto un mese prima delle elezioni amministrative.

vi siete accorti di aver perso le elezioni, ma state continuando su questa strada. Ovviamente noi siamo orgogliosi di come sono andate le elezioni, perché mettiamo un punto per farvi capire come siete sempre uguali a voi stessi, come siete semplicemente dei conservatori.

si dice che le spiagge in Italia sono tante e poiché sono tante, tantissime, non sono un bene limitato, ricollegandosi quindi alla famosa "direttiva Bolkestein", della quale stiamo parlando.

eredità. Dovremmo capire che i beni di cui stiamo parlando sono della collettività, sono beni di tutti, e non è possibile tenere bloccato un settore. Credo che gli stessi imprenditori balneari siano disposti a fare le gare. Ho letto delle interviste nelle quali costoro dicono di volerle fare.

la quale su 8.000 chilometri di costa, solo 2.500 sono dati in concessione. Quanto sono pochi! Abbiamo tantissimi chilometri di costa: chiudiamo tutte le spiagge, mettiamo delle belle barriere, così i cittadini che vanno a fare al mare, se non pagano la loro "gabellina".

Dobbiamo tutelare giustamente gli interessi nazionali e va benissimo se facciamo questo. È importante. L'Italia ha tantissime coste e spiagge e dobbiamo evitare che ci siano

La legge del 1993 prevedeva quattro categorie di classificazione; poi, il secondo Governo Prodi ha detto che erano due e

Ci sono realtà - io sono nato a Massa e conosco bene la Versilia - dove c'è una barriera. Lo stesso succede in Emilia-Romagna e in tanti luoghi dell'Italia. Ieri il senatore Rossi Maurizio parlava della Liguria.

Forse dobbiamo iniziare a fare cose più serie. Dobbiamo dire che in questo Paese le gare si fanno perché, come è stato ricordato anche in questa Assemblea, le gare non ci piace farle. Abbiamo prorogato le concessioni autostradali. Ricordiamoci i concessionari autostradali che pagano il 2,4 per cento dell'introito netto.

Poi dobbiamo capire forse come trovare un modo anche per tutelare le giuste richieste dei balneari, quando sono giuste.

Signora Presidente, credo si debba ristabilire un po' di verità sulla questione dei balneari. Noi non abbiamo accettato la riformulazione, perché riteniamo che la proroga per queste attività debba avere un tempo definito che abbiamo ipotizzato in trent'anni, ma il Governo si è dichiarato contrario, preferendo formule fumose che altri hanno accettato. Senatrice Granaiola, quella formula fumosa la discuteremo con le assemblee di categoria, che lei come me frequenta, e alla fine non potrete raccontare che c'è un adeguato termine. Non c'è alcuna certezza per questi operatori. Non vogliamo difendere privilegi né interessi di casta, perché è chiaro che i litorali restano di pubblica proprietà, ma il problema principale di questa procedura europea, rispetto all'applicazione della "direttiva Bolkestein", è che noi di beni demaniali costieri ne abbiamo tanti e potrebbero essere messi a gara per nuovi operatori. Quindi, si potrebbe consentire a nuovi soggetti di accedervi con delle procedure di gara, vista l'esistenza di molti litorali che potrebbero essere meglio gestiti con attività produttive.

sono stati massacrati. Quindi va bene la lotta all'illegalità, ma non la lotta a un settore produttivo. La storia è abbastanza lunga, ma la ripercorro in sintesi: abbiamo votato

salvaguardare l'ambiente e le imprese balneari per cercare di convincere l'Europa affinché un principio astratto di concorrenza, che riguardi dei beni e non dei servizi, non fosse applicato in maniera ottusa. Infatti, l'Unione Europea è molto contestata anche per il modo astratto e ottuso con cui applica dei principi, perché la concorrenza va garantita,

che possono avere per la Norvegia o per il Nord della Gran Bretagna o per altri Paesi dove le condizioni climatiche non hanno consentito lo sviluppo di un'attività balneare. In questi anni, il

quale inchiesta. Poi Gozi doveva andare in Europa a trattare: figuratevi voi se prendono sul serio Gozi in Europa. Non so se abbia trattato, ma come negoziatore, francamente, forse era meglio mandarci l'ultimo dei bagnini di uno stabilimento balneare, lo avrebbero ricevuto

e forse è andato anche al mare (è di Cuneo e quindi sarà sceso in Liguria per trovarlo); ma comunque gli ho spiegato come stanno le cose, come l'Europa sbagli, come le gare si possano indire per i litorali non occupati da aziende ma che rispettare le imprese è un principio corretto. Non è nemmeno venuto a questo dibattito. Zanetti ha espresso un parere, anzi si è sforzato perché ha detto no ai trent'anni

deve consentire l'accesso al mare anche a chi non paga niente (non ci devono essere muri e barriere) ma non deve essere massacrato o preso in giro come state per fare oggi votando mozioni, che noi non avalleremo, contenenti termini abbastanza generici. E lo fa un Partito Democratico che ha votato la proroga trentennale delle concessioni

dei cittadini che giustamente non vogliono pagare nulla. Spesso sono una specie di immondezzaio, mentre andrebbero gestite e tenute meglio per consentire l'accesso al cittadino che vuole andare con la sua sedia e con il suo asciugamano sulla spiaggia senza dover pagare nulla a nessuno. E allora quelli che sono contro le concessioni,

forse torna in Italia. Ci sono chilometri e chilometri di spiagge che possono essere messi a gara per nuovi operatori, ci sono spiagge libere che gli enti locali dovrebbero gestire meglio, ci sono regole da imporre anche agli operatori privati di accesso e di rispetto dell'ambiente, quindi nessuno vuole la *deregulation* selvaggia; e non si dica che si vogliono rendere le spiagge come la Fontana di Trevi. Basta con queste stupidaggini, perché il litorale rimane proprietà pubblica e ci sono beni che vengono messi a disposizione in cambio di pagamenti che, se necessario, possono essere adeguati e rivisti. La verità è che di fronte alle autostrade il PD si inginocchia e concede le proroghe; di fronte alle piccole e medie aziende italiane preferisce il Per questo non abbiamo accettato il giochino della riformulazione. Infatti, gli imprenditori di quel settore hanno letto l'intervista a «Radio 24» del vice ministro Zanetti e sanno benissimo qual è l'ipocrisia del rito che si consuma oggi, al quale noi non ci associamo perché vogliamo difendere interessi reali e

sarà un problema, perché un'Europa frantumata conterà ancora meno nel mondo e sarà ancora più colonizzata da investitori di altre parti del pianeta. Denuncio l'ottusità europea come un rischio che recherà altri danni all'Europa. Vorrei un'Europa che funzionasse e che avesse maggiore realismo. Colleghi, la Spagna - e che resti agli atti

manteniamo la nostra mozione e la nostra battaglia in difesa di un settore produttivo che è un'eccellenza italiana, che deve essere regolamentato, ma anche rispettato, perché crea occupazione, lavoro e benessere e non è un cancro da combattere e da estirpare. Signora Presidente, noi, a differenza del collega che mi ha preceduto, accettiamo le riformulazioni che il Governo ci ha proposto,

accettati). Riteniamo che il Governo debba fare il possibile per tutelare i nostri piccoli imprenditori dai grandi colossi internazionali. Riteniamo che questo Governo non abbia responsabilità. D'altronde,

in tutti questi anni dai Ministri per i rapporti con il Parlamento dell'uno e dell'altro schieramento. Ricordo a Gasparri che nella scorsa legislatura era un importante Capogruppo di questo Senato e che il suo partito

nella persona del vice ministro Zanetti, per aver accolto la nostra mozione con una leggerissima riformulazione di uno dei vari, numerosi punti che abbiamo posto tra gli impegni

del Gruppo del Partito Democratico e l'ha ricordato, tra gli altri, la collega Granaiola all'inizio della nostra discussione: si tratta di un settore tra i più significativi, peculiari e strategici dell'industria turistica nazionale.

Un settore che ha straordinarie potenzialità in virtù della diffusa presenza sul territorio: 30.000 imprese che arrivano, durante l'estate, a occupare oltre 300.000 addetti. Un settore

che è l'elemento principale dell'iniziativa produttiva di questo settore. A me dispiace che siano prevalsi in alcuni Gruppi - da ultimo nell'intervento del collega Gasparri per il Gruppo di Forza Italia, che egli rappresenta elementi di distinguo su alcuni punti (non su tutti) su cui invece il Senato ha mostrato ampia convergenza. Non a caso, il vice ministro Zanetti ha accolto sostanzialmente tutte le mozioni e gli ordini del giorno presentati, chiedendo evidentemente la riformulazione di alcuni punti. Far prevalere elementi di distinguo - non me ne vorrà il senatore Gasparri che adesso presiede l'Assemblea qualche cedimento anche propagandistico, non aiuta una causa credo largamente condivisa in quest'Assemblea, volta a superare la precarietà e a valorizzare una peculiarità dell'industria turistica nazionale. Ciò nonostante, credo prevalgano gli elementi che fanno concorrere l'intero Senato a invitare il Governo ad una forte iniziativa verso la Commissione europea; settimane, così come ci ha anticipato il vice ministro Zanetti, un provvedimento di indirizzo e di iniziativa legislativa attraverso una legge delega, che, sono certo, recepirà le indicazioni della discussione di queste ore qui in Senato, volta anzitutto - lo dico in maniera sintetica perché il dibattito si è ampiamente soffermato sul merito delle questioni - a definire un percorso di evidenza pubblica e anche di gare per quanto riguarda le nuove concessioni, nello spirito che ci viene richiesto dalla Commissione europea. Questo va fatto individuando criteri assolutamente trasparenti e solidi che, da un lato, possano valorizzare la storia dell'industria balneare italiana (il forte legame con l'ambiente, la diffusione della piccola e media impresa, l'attenzione al mondo del lavoro e alla tutela del mare); dall'altro, evitino un rischio che in larga parte tutti condividiamo, ovvero che l'apertura a procedure di evidenza pubblica, a gare per le nuove concessioni, possa essere il chiavistello per elementi di distorsione del mercato, che tutti vogliamo essere aperto, trasparente, liquido, competitivo, ma che evidentemente non può

l'indicazione che ci viene dalla Commissione europea di superare un regime di proroghe tacite, e quindi di prevedere una sorta di apertura al mercato, nonché tutelare un patrimonio di imprese, di investimenti, di professionalità, di occupazione, di lavoro, che nel corso dei decenni l'industria balneare italiana, del tutto peculiare rispetto ad analoghe esperienze in Europa,

(come se fossimo in presenza di una porta) un'esperienza per aprirne un'altra il giorno dopo, è una metodologia che non farebbe il bene né del mercato,

la mozione che il Gruppo del Partito Democratico ha voluto presentare e su cui il Governo si è espresso favorevolmente - trovare un punto di equilibrio tra questi due elementi: l'apertura al mercato e la tutela e la valorizzazione di un'esperienza di peculiarità del nostro Paese. Per fare questo abbiamo bisogno ancora di tempo. Mi dispiace, senatore Gasparri, che lei abbia indicato nella necessità di definire nelle nostre mozioni un tempo pari a trent'anni un elemento irrinunciabile dell'atto di indirizzo che ha presentato il Gruppo di Forza Italia. Io credo che sia un irrigidimento che che rischia di indebolire un'iniziativa che invece è largamente condivisa da tutti noi. C'è bisogno di tempo non solo per garantire una transizione equilibrata,

tuttora disponibili e liberi, che si può e si deve fare insieme alle Regioni e ai Comuni e per il cui lavoro c'è bisogno di un atto legislativo vincolante, nonché di tempi e di modalità.

del costo dei canoni che le imprese devono pagare allo Stato o comunque alle istituzioni pubbliche, sia anche nella determinazione di chi deve controllare e riscuotere quei canoni. canoni. Penso, non da adesso ma da anni, che sarebbe utile - e questo si può fare anche nella legge delega che il Governo ha annunciato di voler presentare nei prossimi giorni - immaginare una ridefinizione di competenze nella riscossione dei canoni, che io affiderei ad esempio ai Comuni, assegnando loro non solo la riscossione, ma anche la disponibilità di queste risorse. Sarebbe una misura più utile, aiuterebbe le finanze dei nostri Comuni ed avvicinerebbe l'elemento della riscossione in capo alle imprese balneari all'istituzione che dovrà ben gestire quelle risorse, anche con interventi volti a migliorare la tutela dell'ambiente. Di questo c'è bisogno e questo sarà fatto in questo periodo di transizione, che avrà bisogno di tempi adeguati. Un tempo adeguato può essere di pochi anni,

aperta e in una fase in cui credo che commetteremmo un errore se forzassimo scelte e tempi della nostra iniziativa, nel momento in cui c'è un grave contenzioso aperto presso la Corte di giustizia

l'elemento del liberalismo in ognuno di noi, quando non si hanno chiari gli interessi in campo e la necessità di tutelare un equilibrio. Noi abbiamo la necessità di tutelare l'elemento del mercato con l'elemento della peculiarità dell'industria balneare italiana. Sono un po' sorpreso dai toni del Movimento 5 Stelle qui in Senato e del senatore Cioffi, cui affido sentimenti di grande simpatia personale. Non ho trovato traccia di

che si sono espressi durante la campagna elettorale - ad esempio a Ostia - ha usato i toni e gli argomenti da lei usati qui, ma vivaddio la coerenza in campagna elettorale spesso è difficile da trovare. *(Commenti quindi l'apertura a una nuova idea di mercato da parte del Movimento 5 Stelle. Crediamo che quell'idea debba essere misurata con l'interesse generale a valorizzare il patrimonio dell'industria balneare italiana e la nostra mozione va esattamente in questa direzione.

secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni. Dopo la votazione delle mozioni, ai sensi dell'articolo 160 del Regolamento,

Presidente, giungiamo a discutere le mozioni su iniziative contro la corruzione negli appalti nelle grandi opere pubbliche Ha facoltà di parlare il senatore Cappelletti per illustrare la mozione n. 293 (testo 3). *(Brusio).*

Mi chiedo perché ci sia stata tutta questa difficoltà per discutere una mozione che affronta il più grave caso di corruzione mai avvenuto nella storia della Repubblica italiana. *(Applausi sembrerebbe proprio che, come abbiamo visto recentemente per il Daspo per i corrotti, in quest'Aula non si possa e non si voglia parlare di corruzione e, soprattutto, di strumenti efficaci per contrastarla; quantomeno non ne vogliono parlare la maggioranza e una parte di opposizione connivente. Sembrerebbe proprio, signor Presidente, che non si possa e non si voglia parlare di episodi corruttivi che coinvolgono la politica e i suoi più alti livelli, soprattutto se si tratta di episodi corruttivi giganteschi, pervasivi e *bipartisan* che hanno coinvolto tanto il Partito Democratico quanto Forza Italia, tanto le forze di maggioranza quanto quelle di opposizione, come è accaduto nel caso del MOSE.

hanno ricoperto pluriennali ruoli strategici proprio nel Consorzio Venezia nuova, centro di una vera e propria associazione a delinquere, come se non parlare dello scandalo di tangenti più grave della storia della Repubblica italiana sia, in fondo, un modo perché i cittadini possano dimenticarlo più in fretta e non arrivino a imputare anche delle responsabilità politiche, oltre a quelle di ordine penale di competenza delle procure. procure. Colleghi, di fronte a una corruzione che brucia svariati miliardi di euro di risorse pubbliche in un'unica opera non ci sono solo responsabilità penali, ma anche e soprattutto responsabilità di responsabilità di una politica incapace di prevenire eventi corruttivi che, al contrario, hanno praticamente viziato ogni grande opera pubblica realizzata Signor Presidente, lo scandalo del MOSE in Veneto ha messo d'accordo tutti. Si tratta di uno scandalo che ha coinvolto amministratori pubblici, funzionari e uomini politici ai più alti livelli delle istituzioni imprenditori, uniti in un sodalizio criminale che non conosce precedenti. È arrivato il momento di chiedersi se la scelta di affidare progettazione ed esecuzione di una delle opere pubbliche più costose mai realizzate in Italia ad un unico soggetto, non sia stata fatta proprio per promuovere un ambiente fertile alla corruzione, al finanziamento - legale e illegale - ai partiti, ai candidati, alla politica. Non dovremmo chiederci, insomma, se quelle scelte abbiano agevolato i fatti corruttivi a tutti noti, ma se fossero state specificatamente previste allo scopo.

nel 2001 aveva una previsione di spesa di 750 milioni di euro e oggi è arrivata a superare i 3 miliardi di euro, che non sono ancora sufficienti per concluderla di euro, che non sono ancora sufficienti per concluderla - non nasconda esattamente la stessa logica. È arrivato il momento di chiedersi perché il MOSE venne sottoposto a procedura di valutazione d'impatto ambientale con esito negativo e la politica non batté ciglio e come sia stato possibile autorizzare aumenti di costo che hanno portato il valore complessivo dell'opera a quasi 6 miliardi di euro. È arrivato il momento di chiedersi se il carente sistema di vigilanza e controllo delle amministrazioni pubbliche, a partire da quelle ministeriali, non sveli, in tutta la sua gravità, le criticità della legislazione vigente in materia di grandi opere strategiche, e se il tentativo di far scordare in fretta questa vicenda non sia piuttosto funzionale al concedere anche le opere di manutenzione del MOSE agli stessi gruppi imprenditoriali responsabili della corruzione, magari senza gara pubblica, perché ciò sarebbe gravissimo, direi diabolico. Probabilmente una Commissione parlamentare d'inchiesta sarebbe la sede più appropriata per esaminare questi interrogativi, ma la presente mozione, qualora fosse accolta, darebbe un sicuro impulso al ripristino delle condizioni minime necessarie per procedere con l'opera. Per arginare il dilagare dei fenomeni corruttivi, chiediamo in sintesi al Governo che si impegni a procedere all'immediata verifica tecnico-scientifica e contabile del progetto MOSE, avvalendosi di un organismo indipendente e qualificato, composto anche da esperti nel campo della progettazione e modellazione di sistemi marini complessi. alla quale, secondo uno studio del CNR, mezzo milione di tonnellate di cemento, che pesano sui fondali, ha portato

una verifica, al fine di conoscere se il progetto esecutivo abbia confermato i dimensionamenti del progetto definitivo. Chiediamo inoltre al Governo di attivarsi al fine di bandire una gara internazionale per l'espletamento del servizio di manutenzione, inclusa la progettazione e la realizzazione di appositi impianti. poi il Governo ad adottare misure immediate di penalizzazione delle imprese coinvolte nel sistema corruttivo intorno al progetto MOSE e nelle analoghe situazioni che dovessero emergere in relazione ad altre opere strategiche finanziate dallo Stato. Questo si chiama Daspo ed è stato invocato dal Presidente del Consiglio e poi dimenticato. Gruppo M5S)*. Invitiamo inoltre il Governo a riesaminare gli atti e le procedure seguite per la realizzazione delle opere strategiche deliberate o in via di autorizzazione, avviando celermente le conseguenti procedure per il recupero delle risorse sottratte alla collettività attraverso anomali e abominevoli incrementi dei costi di costruzione. e abominevoli incrementi dei costi di costruzione. Invitiamo l'Esecutivo anche a riferire al Parlamento sullo stato delle commesse legate agli appalti per le grandi opere, valutando l'adozione di tutte le opportune iniziative di carattere sia amministrativo sia legislativo volte a consentire la sospensione, la revoca e l'annullamento degli atti e delle procedure viziate da eventi corruttivi. Invitiamo poi il Governo a procedere alla revisione del quadro normativo sull'affidamento dei lavori pubblici, con l'obiettivo prioritario del superamento della legislazione speciale che ha semplificato le procedure in materia di grandi opere derogando la normativa ordinaria e attribuendo poteri immensi ai commissari straordinari. Invitiamo ancora il Governo a provvedere al ripristino delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, disponendo altresì il divieto dell'affidamento di lavori senza gare e senza progetti definitivi, così come il divieto di ricorso a subappalti, nonché ad avviare conseguentemente un processo di revisione della normativa sull'affidamento di lavori e finanza di progetto, al fine di garantire la pubblicità e trasparenza delle procedure ad oggi mancanti. Invitiamo, infine, il Governo a rafforzare la normativa in materia di conflitti di interesse, anche mediante divieti espliciti di contribuzione ai partiti, fondazioni ed esponenti politici da parte di imprese che operano in appalti finanziati con i fondi pubblici, nonché a potenziare, in termini di risorse umane specializzate e di mezzi tecnologici avanzati, gli organismi di vigilanza, monitoraggio e controllo.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, il tema delle grandi opere, della loro progettazione, del loro collaudo e messa in esercizio costituisce da tempo per il nostro Paese un tema spinoso e complesso: spinoso, perché le *performance* che abbiamo registrato negli ultimi anni hanno disvelato spesso un sistema corruttivo e collusivo che ha inciso negativamente non solo sulla credibilità e la buona immagine delle istituzioni pubbliche ma anche sulla perdita di competitività complessiva del nostro sistema Paese; complesso perché la materia degli appalti per le grandi opere pubbliche e la loro progettazione è materia indubbiamente complessa, una materia per addetti ai lavori per antonomasia. E non potrebbe essere altrimenti per grandi opere pubbliche, che spesso si innestano in un territorio di pregio o in contesti ad intenso insediamento urbano o anche, come nel caso del MOSE, in contesti come quello della laguna di Venezia e della sua città di valore inestimabile per l'intera umanità. Un progetto, quello del MOSE, su cui si concentra la prima mozione presentata e alla quale la nostra inevitabilmente si richiama; progetto che, va detto per onestà intellettuale e coerenza politica con il passato, è stato caratterizzato da un'ardita soluzione tecnologica, molto sfidante anche in termini realizzativi e di messa in esercizio, che ha messo e sta mettendo a dura prova la più qualificata ingegneria del nostro Paese. Il sistema MOSE non era l'unica soluzione possibile per ovviare al fenomeno delle maree, ma quella è stata la soluzione intrapresa, anche a fronte di pareri tecnici contrari.

E non meno discutibile è stata la scelta di affidamento al soggetto realizzativo che, come da cattiva tradizione nel nostro Paese, anche in questo caso non è avvenuta per gara, tantomeno sulla base di un progetto esecutivo definitivo asseverato sia dal punto di vista tecnico che sul piano dei costi. Di tutti questi rilevanti aspetti che si sono dipanati nel corso degli anni nella mozione presentata dal gruppo del Partito Democratico viene dato debitamente e oggettivamente conto e a quella rimando per una puntuale ricostruzione, anche storica, delle fasi salienti dell'opera. Singolare anche in questa circostanza è stato il ricorso a strumenti politico-legislativi, tanto per la soluzione progettuale, quanto per la scelta di esperti stranieri per la valutazione degli impatti, quanto ancora per le soluzioni legate all'affidamento realizzativo degli interventi, malgrado pareri contrastanti a livello di procedure amministrative. Ciò nonostante, per correttezza, va anche detto che, pur non essendoci stata una chiara distinzione dei ruoli tra soggetti controllori e controllati (purtroppo anche questa una costante nel nostro Paese, che spesso ha dato luogo a fenomeni distrattivi delle risorse), il progetto nel suo complesso non ha conosciuto significative degenerazioni nei costi. L'incremento dei costi dalla fase progettuale risalente alla fine degli anni Novanta alle più recenti stime, nell'arco temporale quindi di oltre un ventennio, non ha superato il 20 per cento. Per carità, non siamo nel Guinness dei primati nel rigore del rispetto delle stime, ma devo dire che abbiamo avuto in altre circostanze, purtroppo, lievitazioni di costi ben più consistenti per interventi assai meno complessi. Casomai, sarebbe utile conoscere, e lo chiederemo al Governo, dove e per cosa si sono registrati gli incrementi di costi e presumibilmente scopriremmo cose molto interessanti. Ci riserviamo ovviamente di farlo nelle sedi e con gli strumenti più opportuni e non certo con una mozione parlamentare. Ma ci sono due temi di criticità che nella presentazione della nostra mozione non voglio eludere e che tengo invece a rappresentare per alzare il livello di attenzione del Parlamento e sui quali riteniamo di dover impegnare il Governo. Due soli temi a fronte delle molteplici questioni sollevate in altre mozioni, che consideriamo strumentali, non perché infondate, ma per le soluzioni che propongono a fronte di uno stato di avanzamento di circa il 90 per cento dell'intera opera e che rischiano di essere pura demagogia e speculazione politica. Consideriamo per questo irricevibili le proposte di chi avanza la possibilità, adesso, di mettere in discussione la soluzione progettuale e di rescissione dei contratti. E ciò semplicemente perché non si fanno le cose per poi disfarle, specie quando vi sono di mezzo risorse pubbliche, di tutti i cittadini, finalizzate alla soluzione di un problema che non può non essere considerato d'interesse nazionale e non solo di quella comunità. Voglio dirlo con la massima chiarezza, molte delle questioni sollevate e che per noi hanno costituito pregiudizio, sono ormai legate ad una stagione passata, vale a dire quella della legge obiettivo in cui appalti integrati e contraenti generali, nelle dinamiche proprie delle imprese costruttrici, assumevano un ruolo di assoluta predominanza nei confronti delle stazioni appaltanti relegando progettazione e collaudo a fasi subordinate al precipuo interesse dell'impresa. Noi non siamo stati silenti nel passato su questi aspetti. Chi vuole, può andare a vedere gli atti ispettivi che abbiamo presentato nel corso degli anni; ma quella è stata una stagione, come ho più volte avuto occasione di ricordare anche in quest'Aula, in cui una cultura di governo ha avuto un effetto devastante sul ruolo di controllo del soggetto pubblico e in cui i comportamenti degenerativi delle grandi imprese non hanno conosciuto un argine adeguato. Ed è su questo primo aspetto che la mozione reclama in più circostanze un cambio di passo, che in parte sappiamo già essere in corso, ma su cui le istituzioni pubbliche, a partire dalle Commissioni parlamentari competenti, devono essere messe maggiormente al corrente. al corrente. Insomma, noi siamo a questo punto per un più incisivo ruolo di controllo e di vigilanza sull'operato delle imprese in termini di realizzazione e in termini di rendicontazione, prevedendo, come abbiamo scritto, anche la dotazione di organici adeguati nelle competenze e nei numeri del personale della pubblica amministrazione. Un secondo aspetto decisivo per l'effettiva messa in esercizio dell'opera è costituito, in ragione della complessità tecnica dell'opera stessa, semplice nel suo principio di funzionamento meccanico, ma ardita e complessa nel suo efficace controllo delle paratoie, dalla necessità di stabilire l'effettiva congruità delle risorse occorrenti al suo funzionamento e alla sua non banale manutenzione. Su questo secondo aspetto raccomandiamo al Governo davvero la massima attenzione. Il rischio che avvertiamo, nonostante tutti i buoni presupposti, è infatti che il Governo con le sue strutture deputate, rischi di svolgere un mero ruolo di passacarte o si limiti ad un atteggiamento notarile rispetto alle richieste che perverranno dal soggetto gestore dell'opera. Ci permettiamo di suggerire un pieno recupero anche delle competenze allocate nel Consiglio superiore dei lavori pubblici, per un confronto attivo, che vuol dire anche consapevole contrattazione delle risorse pubbliche necessarie al suo costante funzionamento. Il MOSE, come del resto per altri versi il Ponte sullo Stretto o la Salerno-Reggio Calabria, non sono per noi demoni da esorcizzare, né tabù da sfatare: sono opere complesse, caratterizzate da soluzioni ardite, che possono rappresentare la grandezza di un Paese e il suo genio nel mondo - come per secoli avvenuto nel nostro Paese - o possono essere causa di dileggio internazionale e di sperpero di ingente denaro pubblico. Per quanto ci riguarda, non è in discussione la loro utilità e il loro potenziale impatto sull'opinione pubblica internazionale, quanto piuttosto la definizione progettuale degli interventi e le effettive coperture e compatibilità economiche dei relativi piani finanziari. Venezia è una realtà unica al mondo, forse perfino troppo importante nel suo valore storico e artistico per contestualizzarla al solo nostro Paese; merita pertanto che il Governo, qualunque Governo si trovi in carica, senta pienamente il peso delle proprie responsabilità.

nello scrivere questa mozione non abbiamo voluto perdere l'occasione di dare il nostro importante contributo su una questione che ha assillato e, purtroppo - ahimè - continua ad assillare il nostro bel il nostro bel Paese, ossia la corruzione negli appalti nelle grandi opere pubbliche,

dobbiamo essere consapevoli del fatto che abbiamo imprese e professionisti importanti che nel nostro Paese hanno avuto difficoltà nel gestire e realizzare opere

di importanti realizzazioni. Il ragionamento che vorremmo fare è il seguente: il vizio sta nell'uomo, nelle imprese, in chi gestisce o forse nel sistema? Sta nel sistema.

che ha vinto un appalto di una ferrovia che collega il nostro Paese con un Paese confinante. Nel Paese confinante la stessa impresa, partendo con un cantiere unico, è riuscita a terminare

è ancora in fase di cantiere (siamo in ritardo di tre anni e mezzo). È allora appurato che non è stata colpa dell'impresa, ma del sistema. Tornando

tranvia di Firenze che non ci azzecca niente con le opere strategiche. Vorrei veramente un Paese in cui ci fosse una pianificazione seria per quanto riguarda le infrastrutture importanti che devono essere realizzate. Con la mozione n. 585 cerchiamo di dare un nostro modesto contributo, perché a complemento di queste opere ci siano le condizioni affinché il genere umano, cioè i professionisti e le imprese, possano lavorare serenamente e dignitosamente e raggiungere gli obiettivi che sono che sono capaci di raggiungere. Questo è l'importante, su questo dobbiamo focalizzarci e non cercare un pretesto per dire che le grandi opere sono comunque la concentrazione del malaffare. Non è vero; la concentrazione del malaffare

credo che sia un altro momento, un altro mondo e un'altra questione. Qui dobbiamo essere capaci di stare al passo con l'Europa. Mi stupisco di

inopportuno insistere ancora sulla legge obiettivo. La legge obiettivo in questo Paese sappiamo perché è stata realizzata: è nata con un buon intento ma è finita male. Non è più prevista, è stata cancellata; a dire il vero è stata cancellata da Renzi alla sua maniera, per cui nella maniera sbagliata, anche se posso solo dire che sono d'accordo sul fatto che sia stata cancellata.

nell'ambito delle procedure conoscitive per l'approfondimento, la correzione e l'implementazione del decreto legislativo n. 50 del 2016, vale a dire la riforma del codice degli appalti. Per essere chiari, signor Vice Ministro - nel corso di un *question time* l'ho chiesto

Speriamo che il Governo, questa volta, contrariamente a ciò che è stato fatto precedentemente nel corso della seconda lettura al Senato, tenga veramente in considerazione il lavoro delle Commissioni che viene svolto con criterio e giudizio anche da parte delle opposizioni, in

nell'ansia riformatrice che ha colto questo Paese negli ultimi trent'anni (qualche volta mi viene voglia di dire basta con le riforme, perché ogni volta che ne facciamo una sembra che funzioni peggio)

delle richieste di intervento della magistratura ordinaria, in modo particolare delle procure della Repubblica. Si è inoltre sviluppato in maniera abnorme l'interessamento verso uno dei reati tipici relativi all'amministrazione, quello dell'abuso d'ufficio. In molti casi, l'abuso d'ufficio è determinato dal mancato rispetto delle procedure di legge nell'adozione della decisione. Cosa abbiamo ottenuto con questo? Una buona fetta di amministratori onesti, obbligati in molte circostanze ad assumere decisioni con tempestività e velocità, sono incorsi in questo reato, sono diventati oggetto di una critica sociale pesantissima hanno fermato - bloccato in molti casi - le procedure in essere per la realizzazione dell'opera; inoltre determinati danni pesanti nell'attività amministrativa e si è sviluppato un contenzioso oneroso per l'amministrazione pubblica e le casse dello Stato. Penso che sia venuto il tempo di fare una riflessione sui controlli preventivi di legittimità, magari segnando il confine, il perimetro entro il quale tale attività di controllo deve essere svolta, segnando

spettava, per le amministrazioni regionali e per lo Stato, alla Corte dei conti; per i Comuni c'erano i famosi Coreco e Cocico, penso che oggi potremmo individuare nella Corte dei conti, potenziata, di questa attività di aiuto e di contributo a chi amministra la cosa pubblica, affinché non incorra in errore. Infatti, il controllo preventivo, che è un occhio in più, fatto nel momento in cui si forma la decisione e si realizza l'atto sulla base del quale vi è la risposta dei soggetti economici e sociali interessati a quell'intervento,

una riduzione notevole della possibilità di commissione di reati, anche di contenuto decisamente più pesante; garantisce di più chi opera nell'amministrazione in buona fede e limita, molto di più, coloro che, invece, vogliono utilizzare la loro funzione per compiere misfatti.

è successo esattamente il contrario. Siamo andati a finire in contenziosi lunghi secoli, di fronte ad un sistema giudiziario ingolfato anche da questo tipo di attenzioni, che bisognava sicuramente porre in essere per evitare che si consumassero reati e che si danneggiassero la pubblica amministrazione e l'interesse collettivo.

ragioniamo sugli effetti della reintroduzione di una modalità di controllo preventivo; definiamo il perimetro degli atti; definiamo chi sono i soggetti; verifichiamo se questo è utile farlo attraverso specifiche convenzioni tra le amministrazioni pubbliche o lasciamolo, al limite, se fosse necessario, alla responsabile volontà delle amministrazioni pubbliche.

È necessario perché così, penso, si accelera la spesa e si evita un aggravio degli oneri a carico della pubblica amministrazione in caso di contenzioso. È necessario, perché così si garantisce il cittadino, con un'osservanza in più rispetto al passato. Nel passato, infatti, il controllo di legittimità era era diventato solo un peso, anche nella interlocuzione che avevano le amministrazioni nei confronti degli organi di controllo, in quanto non si evitava il contenzioso successivo: il soggetto

non possono essere sottoposti ad un ulteriore vaglio da parte di soggetti della magistratura, ma debbono essere considerati, in ragione dell'avvenuta registrazione, come atti perfetti e quindi in grado di dispiegare perfettamente i loro effetti.

Signora Presidente, ovviamente anche il nostro Gruppo è interessato a dare un contributo e vuole impegnare il Governo a tutte le iniziative necessarie contro la corruzione negli appalti delle grandi opere pubbliche. Si parte sempre dal MOSE, questo Modulo sperimentale

la sua laguna dalle acque per proteggere la popolazione. Ha, quindi, funzioni di protezione civile, ma anche di protezione di tutte le realtà economiche esistenti ed è inutile ribadire che fino al 2010 sono state 191 le grandi alluvioni che hanno superato i 110 centimetri e che solamente dal 2010 in poi hanno iniziato ad essere notevolmente ridotte. Il progetto definitivo di questo sistema era stato approvato nel 2002. Si di un'opera necessaria ed il Governo che lo ha realizzato ha fatto un'opera meritoria. Tale progetto definitivo è stato scelto al termine di un lungo *iter* progettuale e decisionale durante il quale il sistema di paratoie alle bocche di porto è stato confrontato con numerose soluzioni alternative. L'opera, rispondendo a precisi vincoli e requisiti, come ho testé detto, assicura la difesa del territorio del territorio e dei suoi abitanti dagli allagamenti; non modifica gli scambi idrici alle bocche di porto; non ha pile intermedie fisse nei canali alle bocche di porto; non interferisce con il paesaggio con il paesaggio né con le attività economiche che si svolgono attraverso le stesse bocche. Essa è in grado di proteggere Venezia e tutta la laguna da maree alte fino a tre metri e da un innalzamento del livello del mare fino a

laguna fu inizialmente affidata al Magistrato alle acque e poi al Consorzio Venezia nuova, in possesso delle competenze tecniche e professionali adeguate a gestire il complesso degli interventi di salvaguardia. salvaguardia. Per assolvere ai propri compiti di concessionario dello Stato per la realizzazione di studi, attività sperimentali, progettazioni e opere, il Consorzio Venezia nuova si è dotato, nel tempo, di una struttura di pianificazione, organizzazione, gestione e controllo dei vari interventi di salvaguardia nelle diverse fasi attuative, fungendo nel contempo, operativamente, da interfaccia con l'amministrazione concedente, da una parte (ex Magistrato alle acque di Venezia, ora Provveditorato interregionale per le opere pubbliche

Il CVN ha seguito, pertanto, lo sviluppo degli interventi, dalla loro definizione nell'ambito della contrattualistica con l'autorità concedente, alla loro progettazione, fino al loro completamento; nel corso degli ultimi anni, il Mose è risultato un importante volano per l'economia nazionale e locale e fonte di occupazione per migliaia di lavoratori, in via diretta e indiretta, soprattutto oggi, quando lo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione del Mose è pari ad oltre l'85 (qualcuno dice addirittura al 90) per cento di quanto programmato. Considerato che la laguna

legislazione speciale per Venezia prevista dalla legge n. 171 del 1973, che ha dichiarato la salvaguardia di Venezia e della sua laguna problema di preminente interesse nazionale; il progetto Mose è un'opera di avanzata complessità dal punto di vista tecnologico e dal punto di vista ingegneristico, di certo paragonabile

alle tre bocche di porto, che separano temporaneamente la laguna dal mare in caso di alta marea. Complessivamente, 78 paratoie divise in 4 schiere:

e la conclusione dell'opera, perché il bambino va lavato, ma non va gettato al posto dell'acqua sporca. A dicembre 2014, l'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) ha proposto la gestione straordinaria del Consorzio, con la nomina

Il primo impegno consiste nell'adottare, nel rispetto di quanto già programmato e di quanto previsto dal Documento di economia e finanza per il 2016, ogni iniziativa necessaria

Venezia nuova, benché in fase di gestione commissariale, per le attività ancora da realizzare al fine del completamento delle opere. Il terzo impegno è quello di prevedere, in vista del completamento dei lavori e della piena funzionalità dell'opera, misure volte a superare

frode e degli illeciti a favorire il potenziamento della collaborazione con l'ANAC, a promuovere, in relazione alla realizzazione di infrastrutture pubbliche e di eventi, ed infine a dotare le amministrazioni pubbliche delle risorse professionali adeguate ad affrontare le problematiche dell'interlocuzione con i progettisti delle opere e ad esercitare il controllo sui lavori. PRESIDENTE.

è da più di vent'anni (si potrebbe dire dai primissimi anni Novanta), vale a dire dalle prime, acute, scioccanti manifestazioni, mediatiche e politiche, degli accadimenti giudiziari che vanno sotto il nome di Tangentopoli, che i termini «corruzione» e «appalti pubblici» vengono accomunati nell'italico immaginario collettivo. Essi quasi si intrecciano, e, nella percezione comune, l'uno, ahimè, richiama l'altro. Non è indice di buona salute sociale, economica e democratica del Paese. Ciò è dovuto, certo, al manifestarsi degli eventi giudiziari e mediatici, ma, a sommesso avviso di chi vi parla, anche ai continui mutamenti giuridici ed ordinamentali. Carlo Cattaneo, il grande pensatore federalista, già nel 1860 sosteneva che «Ogni mutazione di leggi, che non sia un vero miglioramento, è un danno; perché sospende il rapido corso delle transazioni, diffonde una dubbiezza universale, rende insufficienti tutte le cognizioni pratiche, costringe gli uomini a rifar da capo tutti i loro giudizi e calcoli». Queste parole risuonano oggi più che mai attuali, sebbene totalmente ignorate. Nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile scorso, infatti, è stato pubblicato il decreto legislativo n. 50 del 2016, recante il nuovo codice dei contratti pubblici, entrato brutalmente in vigore lo stesso giorno della pubblicazione, senza la previsione di alcun periodo di *vacatio*. L'assenza di un adeguato periodo di metabolizzazione del nuovo testo da parte degli operatori è stato stigmatizzato anche dal Consiglio di nel suo parere e costituirà comprensibilmente l'elemento di maggiore criticità nel breve periodo per l'applicazione della riforma. È una facile profezia, ma c'è di più. Il nuovo codice degli appalti è stato presentato dallo stesso *premier* Matteo Renzi come una riforma storica, che semplifica le procedure e rende certi gli affidamenti, ma dovremmo ricordare al Governo che se per il codice De Lise era previsto un solo regolamento attuativo, ora gli atti attuativi cui il nuovo codice rimanda sono circa una cinquantina, tra regolamenti e linee guida. Non nascondiamoci dietro l'ipocrisia: è un numero impressionante che reca indecisione, precarietà e blocca l'azione politico-amministrativa e delle stazioni appaltanti. In altri termini, si determina la palude, ci si ritrova nelle sabbie mobili. In tal modo, a tutti dai funzionari della pubblica amministrazione al mondo complesso dell'impresa, ai professionisti, tecnici e consulenti, non è dato conoscere le regole del gioco ed è chiaro che ciò rischia di favorire derive di corruttela. Noi Conservatori e Riformisti vorremmo segnalare anche un'altra questione: la sostanziale sopravvivenza delle gare al massimo ribasso, che negli annunci del Governo dovevano andare in soffitta. Eppure, l'articolo 95 delinea uno scenario diverso: il testo prevede che si possa ancora usare il criterio del minor prezzo per i lavori di importo fino ad un milione di euro, vale a dire la maggioranza dei casi: circa otto appalti su dieci. Ma è proprio qui, in questo *range* di importo, che si annidano statisticamente i fenomeni corruttivi che, sempre nelle intenzioni del Governo, si vorrebbero combattere. Ma la vera norma-beffa si trova all'articolo 77 della nuova legge, relativa ai poteri dell'Autorità nazionale anticorruzione Nelle procedure di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione sulla proposta migliore è affidata ad una commissione giudicatrice composta da esperti del settore. Per garantire la massima trasparenza in questo processo, i commissari saranno estratti a sorte da un apposito elenco predisposto dall'ANAC. Questa regola, tuttavia, vale solo per le gare con importi che superano le soglie comunitarie, vale a dire i 5,2 milioni di euro. Se non si supera questa cifra o se gli appalti «non presentano particolare complessità, la stazione appaltante può nominare componenti interni alla stazione appaltante stessa, nel rispetto del principio di rotazione». Insomma, i commissari saranno scelti dallo stesso ente che assegna l'appalto. Risultato: il 95 per cento degli appalti verrà assegnato esattamente come prima o peggio di prima, con meno trasparenza e

dottor Davigo, che in diverse interviste fa notare come l'Autorità nazionale anticorruzione non sia in grado, né possa sostituirsi alla magistratura ordinaria. Sostenere che sia l'Autorità nazionale anticorruzione a dover combattere il fenomeno corruttivo significa, nella migliore delle ipotesi, millantare un potere che l'ANAC non può avere, mentre nella maggior parte dei casi è sintomo di «ignoranza costituzionale». vorrei far riferimento alla riforma della pubblica amministrazione che il Governo tanto sbandiera come una rivoluzione copernicana, ma che rischia di essere solo uno specchietto per le allodole. Al riguardo, basti prendere atto che il Governo, così come è già successo anni fa con l'abolizione dei Coreco, prevede l'abolizione dei segretari comunali, selezionati all'esito di un lungo e complesso *iter* concorsuale, che sono, invero, i garanti della legalità e i responsabili dell'anticorruzione in tutti gli enti locali. È a questi servitori dello Stato che spetta garantire la conformità, e non solo la legalità, dell'azione amministrativa ed è loro compito rendere più efficace ed efficiente il procedimento amministrativo, riducendo al minimo il rischio di vizi di illegittimità degli atti. Ci chiediamo, pertanto, come la decisione di sopprimere la figura e il ruolo dei segretari comunali possa essere coerente con un'efficace lotta alla corruzione. Avviandomi alla conclusione, signora Presidente, noi Conservatori e Riformisti chiediamo con forza di effettuare una ricognizione dell'attività sino ad oggi svolta dall'ANAC, riferendo al Parlamento al fine di formulare le opportune soluzioni normative e regolamentari atte a rimuovere ogni elemento di incertezza in ordine ai poteri dell'Autorità stessa. Chiediamo, inoltre, di adottare le necessarie modifiche al nuovo codice degli appalti a seguito degli esiti delle attività conoscitive in programma presso le Commissioni parlamentari per l'approfondimento, la correzione e l'implementazione del decreto legislativo n. 50 del 2016. Infine, ma non ultimo per importanza, chiediamo al Governo di valutare

al termine di una tornata elettorale che ha confermato che le priorità dei cittadini italiani non sono le grandi, straordinarie e fantasmagoriche opere tipiche della politica che fino ad oggi ci ha governato. È molto importante, ad esempio, quello che è successo nella città di Roma e quello che hanno detto i cittadini. Si tratta di una città in costante emergenza, in cui continuamente si è cercato di parlare delle se organizzarle o no: il candidato del PD lo ha fatto continuamente e tutta la stampa lo ha seguito allegramente, per quanto sia evidente a chiunque viva in questa città che il vero problema non sono le Olimpiadi e che sono ben altri i problemi che bisogna affrontare. Il problema non sono queste grandi opere.

Che succede in Italia? In Italia abbiamo un bilancio molto interessante a proposito delle grandi opere: le opere previste nella famosa legge obiettivo sono state completate per l'8,3 per cento del totale. Ricordiamo che la legge obiettivo fu voluta da quel grand'uomo e gran ministro del Governo Berlusconi, che era il ministro Lunardi. Tutti noi sappiamo che molte delle opere previste nella legge obiettivo prevedono tante gallerie, stranamente progettate dalla società Rocksoil dello stesso ministro Lunardi. Molte opere - il 57 per cento - sono ancora in fase di progettazione

Sempre negli Stati Uniti, Obama ha stanziato 305 milioni di dollari per finanziare le attività di un organo di vigilanza in materia. Si tratta di una piccola somma, che però ha portato ad

e, ovviamente, alla Salerno-Reggio Calabria, opera che inizia sempre e non finisce mai, anche se mi sembra sia stata inaugurata molte volte. Non sappiamo precisamente quale sia il costo della corruzione, ma sappiamo che l'ordine di grandezza è di decine di miliardi. Ma il costo della corruzione non è solo il costo economico, bensì anche il costo legato all'inefficienza,

nel 2001 erano pari a 3,7; nel 2013 siamo arrivati a 5 miliardi; nel 2014 a 5,2 miliardi e ci sono ancora 226 milioni di euro da spendere. Si doveva completare l'opera nel 2016 e arriviamo al 2018, quando finiremo? Non finiremo mai?

persone a vario titolo coinvolte, come l'ex Sindaco di Venezia, accusato di finanziamento illecito, l'ex presidente della Regione Veneto Galan, accusato di corruzione, l'assessore regionale alle infrastrutture nel 2000 Chisso, accusato di corruzione.

bisogna partecipare. In questo caso non conta vincere ma partecipare, perché magari qualcosa poi ti cade in tasca. Per carità, bisognerebbe essere intellettualmente onesti. Se sei intellettualmente onesto, sei onesto anche nelle altre cose. È un problema di onestà intellettuale. Quando sei chiamato a rappresentare le persone devi sentire dentro di te l'insieme di quelle persone che dicono: fai il nostro bene. Questo bisognerebbe fare, ma questo non succede. Abbiamo provato, come Movimento 5 Stelle, a dire delle cose. Abbiamo prodotto un documento riassuntivo, chiamato Carta dell'onestà, per i corrotti, gli agenti sotto copertura, l'interruzione della prescrizione al termine del primo grado, l'abbassamento delle soglie per i reati finanziari di evasione, il potenziamento del reato di autoriciclaggio, l'innalzamento delle pene per il voto di scambio politico mafioso, lo *stop* alla corruzione negli appalti pubblici, l'abolizione del finanziamento ai partiti, partiti, la revisione del terzo settore, e la *class action*. Noi stiamo sempre a discutere di questo. Discutiamo nelle piazze, continuamente, e poi andiamo a discutere della cosiddetta riforma costituzionale. Sembra che non c'entri e invece c'entra. C'entra quando vediamo, che

di voi non ci possiamo assolutamente fidare. Non dobbiamo pensare che le grandi opere in questo Paese non bisogna assolutamente farle; forse qualcuna bisognerà farla, però dobbiamo vedere quali sono i piani economici e finanziari per far sì che si spendano bene i soldi. Abbiamo presentato una proposta di legge, nella quale chiediamo di prendere tutte le opere della ex legge

Quindi dobbiamo fare le cose che servono e alla gente servono le cose normali, servono le piccole opere che fanno vivere meglio, non le grandi opere! A cosa servono quelle grandi opere? Signora Presidente, la nostra mozione ancora volta vuole mettere al centro proprio questo: vuole mettere al centro l'interesse collettivo, l'interesse delle persone e non l'interesse dei soliti potenti. Hanno già avuto, se ne vadano via questi soliti potenti. Diamo qualcosa alle persone che hanno bisogno che lo Stato intervenga per loro! ho chiesto di intervenire a questo proposito nell'ambito di una serie di mozioni che riguardano di per sé iniziative contro la corruzione negli negli appalti e nelle grandi opere pubbliche, in quanto in almeno un paio di queste mozioni si fa riferimento specifico, anche se forse *incidenter tantum*, alla vicenda del MOSE e al Consorzio Venezia nuova. Il MOSE è una cosiddetta grande opera starebbe per giungere a conclusione, secondo le ultime dichiarazioni ufficiali che prevedono l'ultimazione dei lavori nel 2018. Si tratta di una grande opera ideata per difendere Venezia dalle acque alte eccezionali, anche se va ricordato in questo ambito che le acque alte ordinarie non saranno assolutamente bloccate, nel senso che la zona centrale, ad esempio Piazza San Marco e tutto il vicino centro storico, a 80 centimetri va già sotto e continuerà ad andare sotto l'acqua, perché il MOSE, quand'anche entrasse in funzione, chiuderebbe le proprie paratoie oltre i 110 centimetri. La soluzione MOSE si inquadra nel rapporto che Venezia ha con le acque alte che la inondano periodicamente, e questo fenomeno ha assunto rilevanza nazionale ed internazionale dopo la catastrofica mareggiata del novembre 1966 che aveva completamente sommerso Venezia e gli altri centri abitati lagunari con una marea di centimetri 194 sul livello medio del

all'insieme, o quasi a tutto l'insieme, della società veneziana, comprese associazioni culturali, partiti, patriarcato. Era certamente una grande mangiatoia criminale per quanto riguarda

che la politica faccia in modo che non torni ad essere una mangiatoia con modalità criminali, come rischia tra l'altro, lo dico *incidenter*, di rivelarci e dimostrarci anche la questione delle grandi navi da crociera che continuano a passare all'interno del bacino di San Marco. Nel corso degli anni la storia del MOSE e del Consorzio Venezia nuova è stata caratterizzata da numerose e autorevoli critiche, tutte strumentalmente ignorate per una sorta di autoreferenzialità del Magistrato alle acque di Venezia e del concessionario Consorzio Venezia nuova, concessionario unico, istituto giuridico bandito dall'Unione europea e che ha ancora una vigenza solo qui in Italia. Magistrato alle acque e il Consorzio Venezia nuova non hanno mai voluto rapportarsi seriamente ad alcun confronto tecnico-scientifico sul merito delle argomentazioni critiche sollevate. il risultato che a tutt'oggi, ad opera quasi ultimata, permangono pesanti dubbi sulla sua funzionalità e sicurezza. È solo di due giorni fa l'allarme lanciato da uno dei maggiori esperti, delle maggiori autorità idrauliche del mondo scientifico, il professor D'Alpaos dell'Università di Padova, secondo il quale i lavori del MOSE hanno trasformato la laguna e cambiato le correnti aumentando la velocità dell'acqua e l'erosione, a volte modificando la direzione delle maree, tanto da fargli dire, con riferimento al MOSE: «opera che offende l'intelligenza umana». Ma al di là di queste considerazioni, va sottolineato che, ancora di recente, recentissimi studi del CNR hanno messo in evidenza che si stanno verificando significativi fenomeni di subsidenza in corrispondenza delle opere poste alle bocche di porto, che potrebbero riflettere dei cedimenti differenziali con gravi ripercussioni sulla funzionalità dell'intera schiera di paratoie.

Quando c'è stato il parere per la valutazione di impatto ambientale (VIA) nel dicembre del 1998 si parlava espressamente di un parere negativo, a conferma del precedente negativo parere rilasciato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. A dispetto di questi pareri contrari, si è proceduto come nulla fosse, nel senso che manca ancora quella che chiamiamo ricostruzione storica e, soprattutto, non si è avvertita la necessità di verificare i vari momenti criminali di corruttela che hanno intersecato la storia del MOSE in tutte le fasi decisionali, in particolare accertando - com'era necessario - se le corruzioni fossero non solo utili ad accumulare fondi neri per illeciti finanziari, ma anche indispensabili per l'avanzamento delle varie fasi di un progetto di indimostrata efficacia e di intrinseca instabilità. Non è probabilmente questa la sede più adatta per scendere troppo nel particolare e nel tecnico. Per cui, mi riservo di presentare un'articolata interrogazione in questo senso che tenga conto delle improprietà relative al progetto. di criticità: che l'affidamento della progettazione e dell'esecuzione delle opere è avvenuto a trattativa privata, senza gara e senza confronto tecnico ed economico tra varie e possibili soluzioni. Le opere attualmente in esecuzione sono sostanzialmente diverse da quelle originarie dello studio di fattibilità approvato nel 1982 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per la drastica riduzione dei restringimenti fissi, non garantendosi in questo modo il migliore regime idraulico. Le autorizzazioni politiche non hanno tenuto conto - come dicevo - dei pareri negativi sul progetto di massima del 1990 del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della commissione VIA del Ministero dell'ambiente. Inoltre, le opere complementari, bocciate nel progetto di massima nel 1990 e non presenti nel progetto preliminare del 1994, sono state aggiunte nel progetto definitivo del 2002 e realizzate senza alcuna approvazione dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Si sono poi avviati i cantieri senza aver prima attuato le pregiudiziali sperimentazioni di aumento delle resistenze idrauliche alle bocche di porto (restringimenti fissi), richieste dal Comune di Venezia e dal "Comitatone". È confermata una difficile compatibilità tra il sistema MOSE e lo sviluppo della portualità veneziana. Manca ogni precauzione verso i livelli eustatici, anche in considerazione di quanto valutato dalla Conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici. Inoltre, fenomeni di assestamento dei suoli e delle sovrastrutture a breve e lungo termine comportano effetti sulla sicurezza e funzionalità del sistema per tutta la vita operativa. A questo punto si dovrebbe chiedere cosa fare, perché certamente sono stati spesi molti soldi, ma ancora molti altri dovranno essere spesi. Se continuiamo a tenere conto degli studi e degli accertamenti più recenti, le perplessità non possono che aumentare. Ricordo - ad esempio - che, in materia di criticità strutturale e di comportamento dinamico dell'opera, andrebbe fugato ogni dubbio, considerando che molto di recente, in uno studio eseguito dalla società francese Principia si dimostrava che le paratoie del MOSE presentano fenomeni di risonanza, ovvero sono instabili dinamicamente, soprattutto nei casi di mare agitato.

tecnico, scientifico, autonomo e indipendente debba essere fatto e sia ancora possibile fare. Consideriamo che le risorse necessarie per il MOSE, per la gestione e la manutenzione ordinaria annualmente si aggireranno tra gli 80 e i 100 milioni di euro.

va detto che una valutazione più attenta debba essere fatta con particolare riguardo al comportamento dinamico delle paratoie, delle resistenze idrauliche alle bocche di porto, dei livelli eustatici e dei fenomeni di risonanza. verrà formulata nella speranza che, da parte del Senato e in particolare del Governo, un consenso possa essere dato per tentare di fugare questi dubbi

delle misure di contrasto alla corruzione e per la trasparenza nei grandi lavori e nei lavori pubblici, è già stato realizzato da parte del Governo.

ricordo che già l'ANAC è dotata di poteri e funzioni che il codice raccoglie e disciplina con una certa precisione: in modo particolare per la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le centrali di committenza, nella gestione e nel governo della banca dati nazionale dei contratti pubblici e del casellario informatico, oltre che per tutta la parte riguardante le sanzioni amministrative e pecuniarie nei confronti sia dei soggetti che rifiutano o omettono senza giustificato motivo di fornire le informazioni previste, sia degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta delle stazioni appaltanti o dell'ente aggiudicatore. E segnalo soltanto una parte significativa, ma non definitiva, delle attività che l'ANAC svolge. Ricordo volentieri che il Governo è impegnato a migliorare la qualità delle norme, a ridisegnare i processi decisionali e attuativi delle opere pubbliche, e non soltanto nel nome della trasparenza e della lotta alla corruzione

che consente di perimetrare l'attività del codice, apportando miglioramenti ed emendamenti. Prima di arrivare

che il codice stesso prevede sia un *project review* sia, per quanto riguarda la relazione tra massimo ribasso e gare tenute secondo criteri di natura diversa, un rapporto decisamente più equilibrato. Infatti è vero, senatore Liuzzi, che, per opere aventi un peso inferiore a un milione di euro, rimane come strada principale, e non come strada maestra, quella del massimo ribasso.

il MOSE è un'opera pubblica realizzata, ad oggi, fino all'85 per cento circa dei lavori che erano stati previsti. Sappiamo quali sono gli obiettivi e le finalità. Il Consorzio Venezia nuova, a seguito dei fatti corruttivi emersi e di indebito condizionamento dell'attività e dell'azione amministrativa, venne commissariato con provvedimento del prefetto di Roma in data 1° dicembre 2014. L'intervento fu del prefetto, la richiesta fu dell'ANAC a conferma della ferma volontà del Governo di adottare misure risolute a protezione della legalità. Ai tre commissari nominati vennero attribuiti immediatamente tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione d'impresa con riferimento alla completa esecuzione della concessione, oltre a funzioni di verifica tecnico-scientifica e contabile del progetto MOSE nella sua integrità; un compito speciale che - come affermato dal presidente dell'ANAC Cantone - persegue un duplice obiettivo: prima di tutto evitare che le doverose indagini della magistratura sui fatti illeciti possano ritardare o impedire la conclusione delle opere pubbliche luogo, impedire che l'esigenza di esecuzione dell'appalto e della concessione possa tradursi nell'attribuzione di un indiretto vantaggio per l'autore dell'illecito il quale potrebbe, appunto, trovarsi nella condizione di conseguire un profitto dalla propria attività criminosa. Alcune importanti decisioni, infatti, sono state assunte in merito al cosiddetto *jack-up*, macchinario sofisticato per la rimozione delle paratoie per consentirne montaggio e manutenzione o, a seguito di specifica verifica amministrativa e contabile, al commissariamento della Comar, impresa consorziata il cui operato è apparso piuttosto opaco. Una delle altre questioni che lega per lo meno un paio delle mozioni presentate riguarda l'operato del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere presso il Ministero dell'interno. Tale organismo - lo segnalo e lo sottolineo - svolge un'attività di prevenzione antimafia per le opere di maggior rilevanza per il Paese, peraltro già ricomprese nel piano per le infrastrutture strategiche. L'organismo opera, in particolare, tramite l'emissione di linee guida a valenza generale e attraverso prescrizioni di protocolli di legalità antimafia poi valutati dal Comitato medesimo. Aggiungo che l'infrastruttura MOSE di Venezia, già pienamente ricadente, come altre opere della stessa natura, nella sfera di applicazione delle linee guida dettate dal Comitato che prima ricordavo, è oggetto di specifica attenzione da parte dello stesso Comitato soprattutto dallo scorso mese di febbraio, allorché la prefettura di Venezia ha comunicato la disponibilità, manifestata dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia e dal Consorzio Venezia nuova, rispettivamente stazione appaltante e concessionario dell'opera, a stipulare un protocollo di legalità sulla base del modello tipo contenuto nella delibera CIPE n. 62 del 2015. Proprio al riguardo, il Comitato, anche in considerazione dell'avvenuto commissariamento del Consorzio, ha esaminato prontamente la questione e nella seduta del 16 marzo scorso ha rappresentato la necessità della stipula del protocollo di legalità nelle forme definite dal modello tipo, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori. Infatti, con il decreto del prefetto di Roma del 22 gennaio scorso, viene disposta l'integrazione delle misure già adottate, con espressa previsione che gli amministratori straordinari - leggo «sono tenuti a determinare preventivamente e ad accantonare in apposito fondo fino all'esito dei giudizi in sede penale gli utili complessivamente conseguiti in esecuzione della convenzione stipulata il 4 ottobre 1991 e successivi atti aggiuntivi e attuativi,

si deve estendere anche agli utili conseguiti dalle imprese consorziate, ponendo di fatto in essere una misura cautelativa nella direzione della - leggo - «penalizzazione delle imprese coinvolte nel sistema corruttivo». Segnalo, infine, che, per quanto riguarda i fenomeni corruttivi connessi all'opera, il Governo si è schierato immediatamente a fianco della magistratura affinché continuasse la sua azione nell'ambito dell'accertamento, della verifica, del contrasto e della repressione di comportamenti contrari alla legalità. Il processo penale è in corso presso il tribunale collegiale di Venezia e ha un calendario di udienze già fissato per il corrente anno. Sulla base di quanto comunicato dal Ministero della giustizia, rimangono da definire le posizioni relative alle responsabilità delle persone giuridiche, di cui devono rispondere le principali società partecipanti al Consorzio Venezia nuova - ricordo che è commissariato - oltre al Consorzio medesimo. È stato chiesto e - sottolineo - ottenuto il sequestro dei beni a carico di alcune di esse. Infine, è stato concesso l'utilizzo della banca dati dell'Agenzia delle entrate. Sul punto relativo al rafforzamento della normativa in materia di conflitto di interessi, è utile segnalare che l'azione di Governo è sempre stata quella di sostenere e incoraggiare i progetti di legge di iniziativa parlamentare. Rilevo, per l'appunto, che la Camera ha approvato

Una motivazione è comune a tutte queste mozioni, pur nella diversità dei contenuti: i lavori - lo ricordo, all'85 per cento ad oggi - devono essere realizzati appieno. Questo è il punto comune che le collega, oltre oltre altri tre punti significativi leggibili all'interno dell'articolato. In ultimo, sulla mozione n. 599, presentata dalla senatrice Bonfrisco

l'ennesima occasione perduta dal nostro Paese per dotarci di infrastrutture e non cadere nella trappola della corruzione. Da oltre vent'anni, se non dai primissimi anni Novanta,

- è un grande peccato per il nostro Paese - perché si intrecciano nella percezione comune e finiscono per essere liquidati, poi,

alla fine, concluso il percorso dei vari dibattimenti e processi, si riducono a ben poca cosa. Il cittadino, quindi, ha un doppio danno da tutta la vicenda.

che, per me, sintetizza molto bene il valore del lavoro svolto dal Parlamento, che va sempre collocato nel suo contesto reale.

ogni mutazione di leggi, che non sia un vero miglioramento, è un danno, perché sospende il rapido corso delle transazioni, diffonde una dubbiezza universale, rende insufficienti tutte le

entrato rapidamente in vigore lo stesso giorno della pubblicazione, senza la previsione di alcun periodo di *vacatio legis*, renda la certezza del diritto una chimera e aumenti inevitabilmente il contenzioso, consentendo l'incremento del fenomeno corruttivo in danno degli amministratori della cosa pubblica. Ecco come una legge non correttamente scritta, che non riesce a prevedere tutto ciò che deve poter prevedere nella sua applicazione, anche la parte transitoria, invece che invece che dissipare le nubi della corruzione finisce per alimentare fenomeni corruttivi. Gli italiani conoscono bene l'elenco delle grandi opere rimaste incompiute nel nostro Paese, come i fatti di corruzione negli appalti pubblici, di cui Mafia Capitale è solo l'ultimo capitolo. È del tutto inutile parlare di quelle opere che, ritenute necessarie per lo sviluppo, vennero programmate con tempi di realizzazione e costi ragionevoli, ma che, dopo decenni, sono monumenti incompiuti allo sperpero di denaro pubblico e alla corruzione, nonostante le regole atte a prevenire che i costi di realizzazione lievitassero all'infinito, alimentando la corruzione e i fenomeni criminosi. Noi consideriamo che la maggior parte dei fenomeni corruttivi si annidi nelle gare al massimo ribasso, che in teoria non avrebbero non avrebbero dovuto essere disciplinate nel nuovo codice degli appalti. Nella realtà, l'articolo 95 delinea uno scenario diverso. Il testo prevede che si possa ancora usare il criterio del minor prezzo per i lavori di importo fino ad 1 milione di euro, vale a dire la maggioranza degli appalti pubblici (otto appalti su dieci riguardano, infatti, opere che stanno sotto quell'importo). L'articolo 77 della nuova legge attribuisce all'Autorità nazionale anticorruzione il compito di predisporre un apposito elenco di commissari che dovranno essere estratti a sorte nel caso in cui la gara abbia importi che superano le soglie comunitarie, vale a dire 5,2 milioni di euro. Se non si supera questa cifra o se gli appalti non presentano particolare complessità, la stazione appaltante può nominare componenti interni alla stazione appaltante stessa, nel rispetto del principio di rotazione. I commissari, pertanto, saranno scelti dallo stesso ente che assegna l'appalto. Questo implicherà che la stragrande maggioranza degli appalti verrà assegnata esattamente come prima, o forse peggio di prima, e con minore trasparenza. Ritenuto che l'Autorità nazionale anticorruzione - come molte espressioni della magistratura hanno già sottolineato in diverse occasioni occasioni - non è in grado e non può sostituirsi alla magistratura ordinaria, il cui compito è definito dalla Costituzione stessa, sostenere che sia l'Autorità nazionale anticorruzione a dover combattere il fenomeno corruttivo nella migliore delle ipotesi è un sogno o millantare un potere che essa non ha. Ecco perché abbiamo chiesto di impegnare il Governo a effettuare una ricognizione sull'attività svolta. L'impressione che abbiamo è che carichiamo addosso all'Autorità nazionale anticorruzione tutta una serie di compiti e di aspettative, anche dal punto di vista politico, che l'Autorità stessa poi non è, non può essere e non sarà in grado di sostenere. È importante che il È importante che il processo di lotta vera alla corruzione appartenga a tutte le istituzioni e, quindi, quell'azione possa essere valutata, non per giudicarla, ma per condividerla con le Commissioni parlamentari, in modo da accompagnare questo percorso che si incarna davvero nel tessuto vivo delle istituzioni, perché possa esserci una una particolare condivisione. Ecco perché abbiamo chiesto al Governo di mettere in moto questo meccanismo, che consente - secondo noi - di poter rafforzare davvero tutti quegli atti a garanzia della piena tutela dell'interesse pubblico, che, oltre a essere un fatto tecnico, è un fatto culturale, del quale abbiamo tanto bisogno. Ringrazio il vice ministro Nencini per aver accolto

linee guida da emanare, perché quelle già adottate non hanno ancora completato il quadro dei provvedimenti attuativi e si è ancora in attesa dell'adozione degli

che la politica, le amministrazioni (cioè l'ente locale) e le imprese hanno fatto veramente sintesi compartecipando al finanziamento: 78 Comuni di una Provincia si sono autotassati per cofinanziare un'opera dello Stato. Questa è una cosa straordinaria che - secondo me - signor Vice Ministro - e lei sa benissimo di cosa sto parlando -possiamo portare anche al di fuori dei confini nazionali.

essendo anche un nostalgico della vecchia politica fatta bene, non posso non ricordare una felice

Sono state fatte con grandi difficoltà, anche tecniche. So di sfondare una porta aperta con il senatore Cioffi, perché chi doveva progettare determinate opere di regimazioni idrauliche a seguito di quella catastrofe, non le trovava scritte sul quaderno delle opere pubbliche. Anzi,

dire che parti del nostro territorio consegnano alla storia di questo Paese virtuosismi e capacità di programmazione e realizzazione e altre parti del territorio magari

Signora Presidente, gentili colleghi, sappiamo tutti che, per svolgere in piena libertà le proprie funzioni, i membri del Parlamento godono di particolari garanzie, dell'articolo 68 della Costituzione. Mi riferisco alle cosiddette immunità parlamentari, che comprendono l'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati e l'inviolabilità. Anche l'assenza di vincolo di mandato è una libertà riconosciuta al parlamentare per svolgere la propria funzione di rappresentante della Nazione. Sappiamo anche che, nel corso del tempo, l'abitudine delle Camere a negare l'autorizzazione a procedere nei confronti dei propri membri ha alimentato una profonda sfiducia nei cittadini e trasformato ai loro occhi un principio antico di democrazia parlamentare in un privilegio di casta. Io faccio parte di quei cittadini che lotta perché i diritti non si trasformino in privilegi e oggi, grazie all'esperienza istituzionale, ho una maggiore consapevolezza di quanto sia importante combattere l'abuso, ma, al tempo stesso, difendere il principio. ho vissuto sulla mia pelle cosa può voler dire fare politica con qualcuno che pretende tu sia vincolata alle sue decisioni perché contrario, a suo dire, all'articolo 67 della Costituzione. Ho fatto questa premessa per affrontare una questione di attualità. questione di attualità. In una forza politica che fa della lotta alla casta la propria bandiera esiste ormai l'abitudine di mettere le sedi politiche dei parlamentari nelle abitazioni di persone che, ad insindacabile giudizio del parlamentare stesso, hanno subito un'ingiunzione un'ingiunzione di sfratto ingiusta. Si utilizza cioè la garanzia dell'inviolabilità del domicilio del parlamentare per proteggere un inquilino e "gabbare" così la decisione di un giudice. Una giustizia alla Zorro, in cui il parlamentare agisce di fatto al di sopra della legge, offrendo una protezione *ad personam*. Poco importa se la persona in questione fa parte del *clan* - magari è un attivista del movimento - o è un cittadino qualsiasi, che la sua storia sia meritevole della nostra piena solidarietà, come nel caso di una famiglia di Scandicci, o non lo sia.

volta a far credere che ci siano dei protettori nel Paese, pronti a difendere coloro che si sentono perseguitati dalla giustizia, dal sistema, da Equitalia. Ma non è forse questo un esempio palese di abuso della garanzia costituzionale in questione e, in quanto tale, una vera e propria manifestazione di privilegio di casta, che vede il parlamentare arrogarsi il diritto, non solo di non rispettare una sentenza, ma perfino di impedire che questa venga resa esecutiva? Cosa direbbero, tali signori nemici della casta, se un simile *escamotage* fosse utilizzato da un parlamentare di un'altra forza politica? Non direbbero forse che si aiutano gli amici degli amici? Non parlerebbero forse persino di comportamento di stampo mafioso? Non ci sono altri modi per difendere un cittadino, magari ricorrendo a quella disobbedienza civile, che certo non si fa scudo del proprio essere parlamentare, ma che stimola le coscienze e attira l'attenzione dell'opinione pubblica? Mi domando quindi, in conclusione, se non è il caso di porre maggiore attenzione su questo utilizzo anomalo dell'inviolabilità del domicilio, sancito dall'articolo 68 della Costituzione, perché il diritto alla casa va garantito, ma non con le occupazioni, siano esse in stile Casa Pound o siano esse in stile parlamentare 5 stelle. Del diritto alla casa si deve occupare soprattutto chi governa i territori: le amministrazioni locali hanno il dovere di rispondere a questa esigenza, nel rispetto della legalità e della giustizia sociale. Roma è sicuramente una buona palestra per dimostrare come risolvere il problema del diritto alla casa. [ROMANI

da parte di chi ritiene gli effetti che deriverebbero dall'ottemperanza contrari alle proprie convinzioni etiche, morali o religiose. Colui che effettua tale scelta viene definito obiettore di coscienza. L'obiettore L'obiettore identifica l'interruzione volontaria di gravidanza come l'omicidio di un bambino e, pertanto, è legittimato a non praticare l'aborto: su questo sono d'accordo. Abortire è però una delle scelte più difficili che una donna possa fare. Non è importante quanto si è convinti: l'interruzione è sempre una decisione non facile e non priva di conseguenze emotive e càpita che, fatta questa scelta, la donna scopra che nella sua città, se non addirittura nella sua Regione, i medici che dovrebbero aiutarla ad intraprendere questo difficile cammino si rifiutino di intervenire, in quanto obiettori di coscienza.

Veniamo all'impossibilità di abortire legalmente a Trapani, a causa del pensionamento dell'unico medico non obiettore. Ritengo che questa sia un'interruzione di pubblico servizio, da parte dell'azienda ospedaliera, che dovrebbe garantire l'attuazione della legge n. approvata ben 38 anni fa come legge dello Stato. Non è scandaloso, sapendo ovviamente da tempo che il medico non obiettore sarebbe andato in pensione, che da parte della direzione sanitaria non si sia preso alcun provvedimento per la sua sostituzione? Questa, alla fine, diventa l'ennesima violenza sulle donne e quel che è peggio è che si tratta di una violenza istituzionale. Purtroppo, anche la relazione del Ministero della salute ha ritenuto che i numeri degli obiettori sono tutto sommato accettabili. Come possiamo affermare questo quando su 94 ospedali con reparti di ostetricia e ginecologia solo 62 effettuano interruzioni volontarie di gravidanza? È normale che ci siano Regioni con oltre il 93 per cento di obiettori? Questo è un valore accettabile? Sono diminuite per caso le interruzioni volontarie di gravidanza? Non sarà forse che ci sono stati più aborti clandestini o tentativi che poi si sono indirizzati alle strutture ospedaliere per interrompere l'emorragia? È per tutti questi motivi che già nel 2013 abbiamo presentato il disegno di legge n. 923, assegnato alle Commissioni giustizia e sanità del Senato, nel quale si chiede che almeno il 70 per cento del personale in servizio non sia obiettore di coscienza.

Signora Presidente, gentili colleghi, vorrei rendervi partecipi di una storia che mi ha coinvolto. È una storia commovente ed impegnativa, anche solo a raccontarla. Lo scorso 28 maggio ricevevo, sulla mia casella di posta del Senato, una lettera da parte di un notaio di Bologna che mi informava di essere stata nominata unica erede di un signore di 64 anni che, alcuni mesi prima, scriveva di suo pugno: «Lascio ogni mio bene, immobile e mobile, alla dottoressa Cattaneo, senatrice a vita, affinché li destini, come meglio crede, alla ricerca scientifica». Con queste parole mi si è spalancata davanti la vita di un signore che non conoscevo: il dottor Franco Fiorini, un signore di Molinella, in provincia di Bologna. Dal suo avvocato nei giorni scorsi sono venuta a conoscenza del fatto che il dottor Franco Fiorini era affetto da poliomielite da quando aveva 9 anni, una malattia che gli aveva causato gravi problemi di deambulazione. Nonostante questo, grazie all'affetto e alla protezione dei genitori, era riuscito a laurearsi e ad acquisire anche una posizione dirigenziale in un'azienda della sua zona. condotto una vita piuttosto solitaria, appunto per sua scelta, come conseguenza di questa malattia. Colpisce pensare che Franco probabilmente sia stato tra gli ultimi cittadini italiani a ammalarsi di poliomielite, e colpisce pensare che sia stata solo una manciata di anni a fare la differenza tra un vaccino che, somministrato, avrebbe azzerato il rischio di malattia e un *virus* che lo ha colpito, portandolo a questa vita solitaria, parsimoniosa, ma sempre piena di dignità e autonoma. La sua casa è piena di libri, oltre 5000. Tanti libri di filosofia, tanti libri di scienza. Era una persona che, comunque, ha mantenuto la sua attenzione e il suo interesse sul mondo. Colpisce davvero che un uomo affetto da poliomielite abbia deciso di pensare agli altri, alle altre malattie. Egli non ha rivendicato una rivincita sulla sua malattia, ma ha lasciato ha lasciato questa eredità appunto per coloro che soffrono di altre malattie e per la ricerca in Italia. Colpisce anche che, nel fare questo gesto, non abbia neanche sentito la necessità di essere ringraziato o di accertarsi che il suo lascito finisse in buone mani. Colleghi, questa è una storia inusuale, di un cittadino italiano, di un piccolo paese d'Italia. È una storia che però si incrocia con quella delle nostre grandi istituzioni, del Parlamento, ricordandoci, forse con una certa poesia, che esse sono un importante riferimento per i cittadini e ricordando anche a noi quanto dobbiamo rendere conto ai cittadini, alle persone come Franco. Personalmente è quello che farò, quindi sto lavorando nel pieno rispetto della sua volontà per investire questo patrimonio anche di ideali e di attenzione nella ricerca pubblica italiana. Questo è un impegno cui intendo dedicarmi insieme a quanti tra voi ritengono che la scienza debba procedere libera da condizionamenti ed efficace nel raggiungere gli obiettivi di conoscenza e salute cui quotidianamente lavoriamo. La mia gratitudine quindi va a Franco, anche a nome anche a nome di quei giovani ricercatori italiani che, ancora non lo sanno, ma beneficeranno della sua attenzione verso la conoscenza e dell'intensità e dell'oculatezza della sua vita. senatrice Cattaneo, per aver portato in quest'Assemblea l'attenzione e il ricordo di una persona così importante, e di aver reso onore, secondo me, alla scelta. La ringrazio anche a nome della Presidenza.

limitate nel tempo per particolari soggetti. Si tratta di un istituto nato negli anni Novanta attraverso un protocollo sulla politica attiva del lavoro e sull'occupazione. Poi ci sono stati dei successivi interventi legislativi, in particolare nel 1994, nel 1996, nel 1997 e così via. di anni, il decreto interministeriale n. 66 del 2001 ha stabilito che i soggetti impegnati in attività di lavoro socialmente utile, riconducibili a funzioni di assistente amministrativo e tecnico nelle istituzioni scolastiche,

È proprio l'antitesi: si parla di stabile occupazione e collaborazione coordinata e continuativa nel 2001, ma queste persone, nell'anno 2016, ancora sono Co.co.co.

che continuino ad essere Co.co.co. a vita.

ha messo la parola fine, perlomeno in questa fase, alla questione lunga, faticosa e problematica del riconoscimento dell'adozione del figlio del *partner* all'interno di coppie dello stesso sesso. È un tema che aveva impegnato questa

chiara che conferma le sentenze che in giro per l'Italia avevano già avuto un'affermazione univoca. Penso alle varie sentenze

dovrà avvenire attraverso il ricorso a un giudice, che dovrà valutare un superiore interesse del minore, esattamente come noi avevamo previsto all'interno della legge sulle unioni civili. C'è solo una differenza tra la nostra proposta e quel diritto che oggi la Cassazione riconosce: noi, nella nostra proposta, avevamo limitato la possibilità di adozione